gestione dei rifiuti, cui risponderà il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Orlando. Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, voglio cogliere quest'occasione per sottoporre un tema che, come Partito Democratico, abbiamo sviluppato in una mozione a prima firma del presidente Zanda, poiché il tema del dissesto idrogeologico si pone oggi come un problema nazionale, non solo regionale, che non può più essere fatto rientrare nella logica dell'emergenza, viste sia la frequenza degli eventi sia la gravità delle conseguenze sui territori coinvolti, connesso com'è anche ai cambiamenti climatici cui siamo sottoposti. Questa logica, signor Ministro, deve essere sostituita da quella della prevenzione e della messa in sicurezza del territorio, uniche vere strade da percorrere anche in vista di un uso intelligente ed efficace delle risorse. Allo stato attuale, invece, quasi tutti gli interventi per la difesa del suolo realizzati nel nostro Paese sono interventi strutturali di difesa passiva che in termini di costo e di efficacia si sono rivelati non pienamente soddisfacenti. Auspichiamo perciò che una moderna strategia di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici e ai rischi si basi, certo, sulle opere, ma limitandole a quelle davvero irrinunciabili, e si indirizzi verso un approccio più in sintonia con i processi naturali, collegando obiettivi di riqualificazione dell'ecosistema fluviale alla diminuzione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico. In quest'ottica abbiamo molto apprezzato l'intervento da lei tenuto in Commissione ambiente sulle linee programmatiche del suo Dicastero, in cui ha messo in rilievo la necessità della riduzione del rischio idrogeologico e il ritorno a una politica attiva Tra gli impegni che spero il Governo accolga, voglio sottolineare, in particolare, l'adozione di politiche che, contrastando il fenomeno dell'abbandono dei terreni, del disboscamento e quindi dell'improduttività del terreno, soprattutto degli Appennini, riconoscano il valore strategico dell'agricoltura come presidio e strumento che favorisce la manutenzione ordinaria del territorio. Per queste ragioni le chiedo, signor Ministro, se e in quali tempi il suo Dicastero intenda predisporre

Signora Presidente, onorevole Ministro, colleghi, oltre 6.000 sono i Comuni italiani in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico, l'82 per cento una fragilità che riguarda parecchie Regioni: Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d'Aosta e la Provincia di Trento, dove ben il 100 per cento dei Comuni è classificato a rischio. La dimensione, tra l'altro, riguarda circa 30.000 chilometri quadrati, quindi all'incirca il 10 per cento del territorio nazionale, e ben 5 milioni di nostri concittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane e alluvioni. Da questi numeri nasce la necessità di riflettere attentamente per sviluppare percorsi risolutivi in grado di rispondere in modo efficace alle ripetute emergenze collegate al rischio idrogeologico nel nostro Paese, emergenze che scattano ormai sistematicamente ad ogni autunno, e non solo, a causa di una mancata adeguata politica di prevenzione e di governo del territorio. In conseguenza di questa premessa, le chiedo quali siano le politiche di prevenzione che lei sta già immaginando sull'intera vicenda. Come pensa il suo Dicastero di affrontare queste probabili, possibili (facciamo gli scongiuri che non ci siano) emergenze? E soprattutto, a quanto ammontano e da dove sono reperibili le risorse necessarie da destinare a questo strategico programma?

Vogliamo sapere dal Ministro se concorda con noi sulla necessità di intraprendere un percorso legislativo volto alla tutela dai danni ambientali derivanti dalle trivellazioni, che - è provato da studi autorevoli e indipendenti - sono connessi con l'alto rischio di sismicità indotta e di inquinamento di terra, aria ed acqua. L'acqua è più preziosa del petrolio e non sostituibile a differenza di quest'ultimo. Quando abbiamo compromesso una falda acquifera abbiamo perso una ricchezza di tutti per sempre. Il petrolio non convenzionale, quello che stiamo cercando «grattando il fondo del barile» non più nelle aree desertiche, ma vicino ai centri abitati su aree di ricarica degli acquiferi (in Basilicata se ne contano ben 8 piattaforme), in zone a noto rischio sismico e ad alto rischio di energia tettonica accumulata oppure a poche centinaia di metri dagli ospedali, il petrolio amaro e pesante ha costi crescenti ed energia netta decrescente con costi ambientali incalcolabili. Il danno evidentemente non deriva solo dall'eventuale incidente, che causerebbe un disastro ambientale certo, ma dall'attività stessa; si provocano danni sin dalle attività ispettive, che si attuano con microesplosioni controllate cui devono seguire segnali riflessi, dannosi alla fauna marina; con i fanghi e fluidi perforanti, che per appesantire, per andare più a fondo a cercare, vengono caricati con sostanze anche molto pericolose, di cui le compagnie non sono tenute a dichiarare la composizione, e attenzione, si legge dalla relazione dell'ENI testualmente che «le perdite sono frequenti», ordinarie, e con lo smaltimento, per un barile si contano ben 10 barili di scarto...

Ci sono stati un morto, numerose famiglie sfollate, centinaia di milioni di euro di danni alle case, alle attività produttive e a beni collettivi come strade e opere idrauliche. C'è un aspetto su cui vorrei conoscere il parere del Ministro dell'ambiente. Uno studio commissionato dalla Regione Veneto ha recentemente confermato l'opportunità e la fattibilità di un canale scolmatore sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, già in gran parte espropriato a fini idraulici, atto a convogliare in laguna parte dell'acqua del Brenta, a partire da Vigonovo a sud-est di Padova. Tale canale avrebbe almeno quattro vantaggi: proteggerebbe i territori di Padova e Vicenza e parte del veneziano dall'esondazione del Brenta e del Bacchiglione, quali le opere a tutt'oggi previste non sono in grado di far fronte in caso di piene simili a quelle del 1966; contrasterebbe i fenomeni erosivi che stanno interessando parte della laguna di Venezia; garantirebbe un sollievo all'agricoltura del veneziano in caso di siccità; potrebbe infine essere un passo importante verso la realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia, economicamente valida in caso di costruzione del porto *offshore* dell'Alto Adriatico. Per la realizzazione dell'opera, che costa fra i 200 e i 300 milioni di euro di euro - meno di un ventesimo del sistema Mose e molto meno dei danni idraulici degli ultimi tre anni nelle sole province di Padova e Vicenza - è possibile anche l'accesso ai fondi europei, ma è necessaria un'azione concordata fra la Regione Veneto e lo Stato.

Signora Presidente, signor Ministro, come già detto, è accertato che oltre l'80 per cento dei Comuni italiani ricade in aree classificate a potenziale rischio idrogeologico. Annualmente, e anche il recente passato ne è stato testimone, si verificano disastri ambientali, frane, smottamenti ed esondazioni con perdite di vite umane e ingenti oneri sociali ed economici. Per questo, signor Ministro, le chiedo quali iniziative urgenti intenda adottare, anche di natura normativa, per realizzare un piano strutturale di finanziamento di interventi contro il rischio idrogeologico e per la difesa del suolo che in primo luogo privilegi la logica della prevenzione rispetto a quello della gestione dell'emergenza; sblocchi le risorse già previste dalla scorsa legislatura dagli accordi di programma sottoscritti con le Regioni per gli interventi prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico; coinvolga gli enti locali e le Regioni per l'attuazione degli interventi; infine, in ordine alle risorse provenienti dallo Stato, dalle Regioni e di quelle proprie degli enti locali, preveda l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno delle spese destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico.

da rischio idrogeologico in forme gravissime, gravi e meno gravi. Purtroppo, solo negli ultimi tre anni lo Stato ha stanziato 1 miliardo di euro per le emergenze causate dal rischio idrogeologico. Per la prevenzione invece sono stati stanziati solo 2 miliardi in 10 anni. Questi dati, signor Ministro, ci dicono che non è più assolutamente rinviabile un piano straordinario

Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, si richiede al Ministro se ritiene opportuno ricostituire la Direzione generale per la difesa del suolo,

un approccio integrato per le problematiche di acqua e suolo, visto che con un apposito decreto l'ex Ministro aveva voluto unificare in un'unica megadirezione le competenze relative a rifiuti, bonifiche, acqua e suolo, affidandone la direzione a persona fra l'altro sprovvista di titoli idonei, come peraltro riconosciuto dalla magistratura ordinaria. Si chiede anche, visto che il Corpo forestale

i costi, dal momento che erano diventati veri e propri «stipendifici», perché non prevedere che tali consorzi vengano ristrutturati con proprie funzioni, al fine di essere utilizzati in modo utile e fattivo per il controllo idrogeologico del territorio italiano? Quindi, signor Ministro, occorre

contiene una disposizione volta a semplificare l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure prescritte dal regolamento n. In particolare, le procedure stabilite in tale decreto sono proporzionate ai materiali da scavo prodotti nell'ambito delle cosiddette grandi opere, mentre esse possono risultare eccessivamente gravose e sproporzionate per quelli prodotti in cantieri di minore entità. Quindi si è ritenuto di limitare l'applicazione delle predette procedure alle attività od opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

di incorrere nelle infrazioni europee e colma i vuoti legislativi che il comma 1 avrebbe determinato, le chiedo se intenda modificare il successivo decreto‑legge n. 69 del 2013, poiché si ritiene che il comma 2‑*bis*, aggiunto all'articolo 184‑*bis* del decreto legislativo n. del 2006 non sia da solo sufficiente a chiarire il regime applicabile alle terre e rocce da scavo al di fuori della fattispecie da esso considerata. Inoltre, poiché il disegno di legge sulle semplificazioni fiscali ed amministrative prevede, tra le altre cose, la semplificazione normativa

Signora Presidente, onorevoli senatori, cercherò di dividere le questioni poste in tre grandi temi (la questione delle risorse; la struttura di intervento, la filiera istituzionale e i soggetti abilitati; le azioni che il Ministero sta promuovendo) provando a dare poi una risposta alle questioni più specifiche che sono state poste. Mi scuserete se lo farò in modo assolutamente schematico, dato il tempo limitato. Vorrei ricordare, come premessa, che il bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del e che fin dall'avvio dei finanziamenti risalenti alla legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo si è verificato quello che rappresenterà poi uno dei problemi ricorrenti, che si è anche ripresentato in questi mesi: la commistione tra i fondi utilizzati per la prevenzione e quelli destinati alla riparazione *post* evento. I fondi inizialmente stanziati, pari a 1.000 milioni di euro, sono stati in parte distolti per far fronte infatti agli eventi calamitosi verificatisi in alcune Regioni italiane e poi azzerati da successive manovre finanziarie. Ad oggi, il valore complessivo degli accordi sottoscritti, considerate le risorse FAS statali destinate dalla legge finanziaria 2010 quale bilancio e messi a disposizione del Ministero e le risorse regionali, è pari a 2.075.000.000 di euro, per oltre 1.500 interventi finanziati, suddivisi in ulteriori stralci funzionali. Il quadro complessivo della situazione contabile degli accordi di programma, al gennaio 2013, rivela che, grazie alle risorse proprie di bilancio, il Ministero dell'ambiente ha potuto erogare ai soggetti attuatori, dal 2010 fino ad oggi, 544 milioni di euro, a fronte di 814 milioni di euro. Tuttavia le Regioni non hanno risposto con pari sollecitudine alla necessità comune di mettere a disposizione le loro risorse, così come concordato in fase di accordi. Anche le problematiche derivanti dal vincolo di Patto di stabilità hanno inciso naturalmente su questo. Infatti, ad una ricognizione effettuata al giugno 2013, risulta che sono state trasferiti sulle contabilità speciali dei commissari complessivamente per tutte le Regioni firmatarie solo 140 milioni di euro, a fronte dei 1.261 destinati dagli accordi stipulati con le Regioni stesse. Inoltre, mentre gli accordi di programma con le Regioni del Centro Sud sono oggi coperti con la delibera CIPE n. 8 del 2012, quelli sottoscritti con le Regioni del Centro-Nord hanno ricevuto sola parziale copertura dalla delibera CIPE n. 6 del 2012. A proposito di questo tema complessivo, quali sono le linee sulle quali credo ci si debba muovere? Una l'ha indicata la senatrice De Petris: individuare i progetti già oggettivamente cantierabili e dare loro priorità. L'altra è la rimodulazione del Patto di stabilità. Si tratta di un tema che va discusso nella sede propria, cioè quella europea, così come anche quello della modulazione dei fondi europei dal 2014. Nell'ultimo Consiglio europeo dedicato all'ambiente, ho sollevato con i rappresentanti di altri Paesi esattamente questo tema: la questione dell'adattamento non può essere esclusivamente posta in di misura di limiti e condizionamenti allo sviluppo, che pure sono assolutamente necessari, ma va anche affrontata in termini concreti per realizzare delle strategie di adattamento. Da questo punto di vista, il dissesto idrogeologico è una delle priorità, soprattutto in aree storicamente sottoposte a questo tipo di fenomeno, come è l'Italia. Il fenomeno non va approcciato semplicemente come in grado di produrre rischi, ma anche come una delle cause dell'aumento del *gap* infrastrutturale del nostro Paese. Non ci sono solo lutti e case che cadono o versanti che franano: ci sono ponti, ferrovie e autostrade danneggiate dal dissesto idrogeologico, ciò che crea un aumento del*gap* dal punto di vista infrastrutturale, mentre si pensa di realizzare nuove opere che dovrebbero colmare questo *deficit* che progressivamente si realizza. È quindi importante che, nella definizione delle misure che avranno l'avvio dal 2014, il tema del dissesto idrogeologico sia al centro dell'attenzione dei decisori a livello europeo e della Commissione, che devo dire in quella sede ha dato un primo riscontro positivo. C'è poi un altro aspetto che credo debba essere adeguatamente affrontato, e riguarda il tema della prevenzione. Da questo punto di vista, il Governo ha giorni fa un provvedimento sul tema del consumo del suolo, che rappresenta un primo passo per dare una risposta strutturale al tema. La sostanza di questo provvedimento è la seguente: si può costruire soltanto se prima si è dimostrato di avere riutilizzato e di essere intervenuti sul patrimonio edilizio esistente. Questo è un principio che, se affermato e rapidamente convertito, anche con il contributo che le Camere potranno dare, può consentire di fare un passo avanti significativo. Aggiungo un altro aspetto che ritengo importante, fondamentale, e che è stato posto in alcune domande: è stato posto in alcune domande: il dissesto idrogeologico, come è stato segnalato, non si contiene esclusivamente con misure di carattere vincolistico e interventi, ma anche con una manutenzione costante del territorio. Da questo punto di vista, il tema dell'intervento sulle aree boscate e nelle aree agricole è assolutamente centrale. Per questo quella legge, che nasce con uno scheletro molto ridotto, può essere sede anche di una serie di interventi a sostegno della manutenzione e della redditività stessa dell'intervento sul bosco ed il suo esame può costituire un'occasione nella quale il Parlamento può contribuire a dare una risposta strutturale a questi temi. Quanto alle filiere istituzionali,

è pur vero, però, che ci sono soggetti che storicamente hanno assunto altre funzioni che possono in parte contribuire ad affrontare il fenomeno. La sollecitazione del senatore Barani rispetto a una

ho da principio manifestato alcuna particolare simpatia verso questa fonte di approvvigionamento contenuta nella strategia energetica nazionale; prima di affermare un nesso causale tra le trivellazioni e i fenomeni sismici credo occorra la pronuncia incontrovertibile di autorità scientifiche. In questo senso mi sono attivato e mi attiverò affinché l'ISPRA si esprima su questo nesso, che credo sia un punto sul quale non si può equivocare. C'è l'esigenza di capire se effettivamente tale nesso esiste e sulla base di questo dare dare valutazioni in ordine alla crescente domanda di trivellazioni, rispetto alla quale attualmente rispondiamo semplicemente considerando due elementi: la distanza dalle coste per quanto riguarda il mare e la contiguità rispetto alle aree protette. Se ci fosse questo ulteriore elemento è chiaro che l'intero quadro normativo dovrebbe mutare, ma questo elemento credo debba essere certificato da autorità scientifiche, che al momento mai hanno prodotto una incontrovertibile valutazione in questa direzione.

del possibile rischio. Un'altra misura che il Ministero sta assumendo è quella della definizione di un fondo per l'abbattimento degli abusi edilizi realizzati in aree di dissesto idrogeologico. Credo sia un segnale importante: esso non ha la pretesa di affrontare complessivamente il tema dell'abusivismo, che merita una sede propria di riflessione e rispetto al quale a mio avviso a mio avviso ci deve essere una indicazione molto netta, che ho già ripetuto in numerose occasioni, ma, per quanto riguarda le realtà nelle quali si combinano contemporaneamente rischio e illecito, credo che lo Stato debba mettere i Comuni nelle condizioni di intervenire, dando una risposta che è anche a tutela dei cittadini. Per quanto riguarda il tema della Direzione e dell'assetto del Ministero sul tema del dissesto idrogeologico, vorrei rispondere in modo organico attuando le indicazioni contenute nella *spending review*, poi integrate da una recente norma

Sulla questione acqua, ho chiesto alle Commissioni competenti di Camera e Senato di definire un atto d'indirizzo in ordine alla produzione

sono realizzati molti inconvenienti in ordine a molti importanti investimenti e anche numerosi abusi, che hanno prodotto danni al nostro territorio. Quindi, sulla base degli elementi contenuti nel disegno di legge, vorrei avviare un confronto, con le Commissioni competenti, per consentire poi, all'approvazione del disegno di legge, di avere una disciplina organica che riguarda il tema delle terre e rocce da scavo. PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per un minuto ciascuno.

ci ha detto su questo tema sono molto importanti e sicuramente, per quanto riguarda il Partito Democratico, troverà, nelle Commissioni di competenza cui ha chiesto un contributo e una mano per l'approvazione di atti di indirizzo su tematiche prioritarie, una forza che proverà a dare il suo contributo. Credo che ci siano punti importanti e qualificanti nell'azione che il suo Dicastero ha indicato, che credo debbano trovare un coinvolgimento importante di tutta la filiera istituzionale: Regioni, Province, Comuni

signor Ministro, i suoi intenti sono sicuramente buoni. Ci ha convinto la risposta in materia di politica di prevenzione. Tra l'altro, è giusta l'intuizione che riguarda l'assetto complessivo del territorio. A tal proposito,

Per quanto riguarda invece il resto delle questioni sollevate, devo chiederle però una maggiore forza e una maggiore incisività, perché è chiaro che bisogna attivare delle politiche per trovare maggiori fondi e maggiori risorse. Per quanto riguarda non solo la mia parte politica, ma credo tutta la Commissione ambiente, saremo sicuramente assieme a lei per portare avanti questa che non è una battaglia, ma è una rivendicazione necessaria nell'interesse del nostro territorio, del nostro Paese. le vorrei dire, riguardo alla risposta che mi ha dato, che la letteratura internazionale purtroppo ha dimostrato invece l'esistenza delle trivellazioni rispetto alla sollecitazione sismica, chiaramente là dove le zolle già sono cariche. Chiaramente, se questo non avviene, non avverrà neanche il terremoto. In particolare, con riferimento al terremoto dell'Oklahoma, la cosa è stata accertata, è stata prolungata nel tempo, ci sono state molte scosse e gli scienziati si sono pronunciati in tal senso. Tra l'altro, devo dire che tutta la documentazione a nostra disposizione è in inglese, perché purtroppo io credo che nel nostro Paese ci sia un grossissimo problema di conflitto di interessi:

all'indipendenza di molti intellettuali, abbiamo anche noi la possibilità di avere dei pareri altri, indipendenti: a questi ci dobbiamo riferire. [DALLA signor Ministro, per il suo intervento. Prendo atto della grande rilevanza da lei data all'idea di passare ad interventi fortemente basati sulla prevenzione.

Signor Ministro, in ordine all'istituzione del fondo per l'abbattimento degli abusi, tutti i Comuni devono essere aiutati a fare azioni di prevenzione, e non solo quei Comuni che non hanno vigilato, consentendo

sul tema dello sblocco del Patto di stabilità. Ovviamente il Gruppo della Lega Nord si dichiarerà soddisfatto quando vedrà concretizzarsi le sue intenzioni. [DE

proprio per la manutenzione delle aree...

MORGONI *(PD)*. Signor Ministro, nelle dichiarazioni programmatiche rese alla Commissione ambiente del Senato, lei ha indicato il tema dei rifiuti come una grande emergenza del nostro Paese. È innegabile che sia così. Solo pochi giorni fa la Commissione europea ha proposto sanzioni per oltre 250.000 euro al giorno (circa 80 milioni di euro annui) a causa delle ripetute inadempienze in materia di gestione dei rifiuti in Campania; in questo senso le chiedo notizia degli interventi in materia di impiantistica in questa stessa Regione. Ma, allargando lo sguardo, possiamo constatare che tra i 27 Paesi dell'Unione europea l'Italia è al ventesimo posto nella classifica per 1'efficienza nella gestione dei rifiuti, dei quali finisce in discarica, contro una media degli altri Paesi pari al 38 per cento. Occorre certo intensificare la raccolta differenziata con vincoli più severi e norme più rigorose, ma soprattutto premiando i comportamenti virtuosi, ciò che è stato sempre annunciato, di fatto mai realizzato, ed oggi palesemente contraddetto dalla TARES. Considerando, però, che l'entità complessiva dei rifiuti risultava ancora in crescita nel 2010, la vera sfida è quella del contenimento attraverso un piano nazionale per la riduzione e la prevenzione degli stessi, come previsto dalla direttiva quadro dei rifiuti. quali tempi preveda per l'approvazione del piano e quali politiche specifiche e strutturali all'interno di esso intende promuovere nei confronti di aziende produttrici, distributrici e associazioni dei consumatori per una efficace azione di contenimento della produzione e dell'utilizzo degli imballaggi, che rappresentano complessivamente il 50 per cento

*(PdL)*. Signor Ministro, la situazione di crisi relativa all'emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti coinvolge almeno quattro Regioni: Lazio, Calabria, Campania e Sicilia, quasi un terzo della popolazione nazionale, grandissime aree metropolitane come Napoli e Palermo. Per quanto riguarda la Regione Lazio, e Roma in particolare, le chiedo quale sia lo stato di efficienza dei sistemi e degli impianti di trattamento attuali, compresi quelli che non sono afferenti alle pubbliche proprietà, quali siano le possibili iniziative utili a colmare il *gap* impiantistico, con particolare riguardo agli impianti per la produzione di energia dal recupero dei rifiuti. Chiedo altresì quali siano le iniziative, promosse dal suo Dicastero, atte a coprire l'eventuale interregno tra la chiusura di Malagrotta e l'apertura del nuovo sito, onde evitare nel prossimo futuro di trovarci nell'analoga, delicata, situazione emergenziale del territorio campano. Chiedo inoltre come intende il Ministero verificare i risultati conseguiti a seguito del recepimento della cosiddetta normativa europea sui rifiuti, con particolare riferimento ai miglioramenti ottenuti in ciascuna delle attività previste dalla gerarchia degli interventi di cui all'articolo 179 del codice ambientale.

Il cuore di tutto questo è che i rifiuti non devono essere mai visti come una risorsa, perché altrimenti andiamo a costruire una società basata sul rifiuto; creiamo una filiera di trattamento che ha continuamente bisogno di produrre rifiuto affinché, in mezzo,

sbagliate. Chiediamo come sia possibile insistere con l'incenerimento dopo che fior di direttive ci dicono di non farlo, e noi sappiamo che dal 2020 non si potrà più ricorrere a questo tipo di strategia. Qualunque impianto di incenerimento ha un tempo di ammortamento ventennale, quindi siamo fuori da ogni logica già nel momento in cui lo incentiviamo. La terza domanda è: in quale modo vogliamo far sì che i produttori diventino responsabili di quello che immettono nel commercio, considerato che finora la responsabilità ricade sull'utente finale (il consumatore si accolla

Signora Presidente, gentile Ministro, il recente decreto ministeriale 20 marzo 2013 ha previsto un progressivo riavvio del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, meglio noto come SISTRI. Il SISTRI rappresenta una pesante eredità. L'istituzione di questo sistema è stata accompagnata fin dall'inizio da dinamiche poco trasparenti relativamente alla rete di operatori coinvolti e ai controlli stabiliti e da pesanti farraginosità operative; criticità che ne hanno rimandato l'attivazione effettiva fino ad oggi, danneggiando altresì quelle aziende che già per gli anni 2010-2011 avevano anticipato il contributo di copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema. Queste problematiche sono state oggetto di miei interventi già nella precedente legislatura, nonché di inchieste giornalistiche che hanno rivelato punti oscuri e presunti illeciti sui quali l'esigenza di chiarimento è alta, a partire dall'opposizione del segreto amministrativo su su progetto, opere, servizi e forniture per la realizzazione del sistema, affidati senza procedure di evidenza pubblica alla Selex Service Management del gruppo Finmeccanica, amministrazione (DigitPA) ha evidenziato come non compatibili col principio di trasparenza. Sono pertanto a chiederle, signor Ministro, quali siano le reali dinamiche che hanno condotto alla nascita e alla struttura del SISTRI, oltre che la natura del contratto intercorso tra il Ministero e Finmeccanica, e quali prospettive vi siano per il futuro in vista della prossima riattivazione auspicata con primo termine al 1° ottobre 2013 in merito alla sopravvivenza del sistema, alla trasparenza delle dinamiche che lo interessano, alle sue eventuali riconfigurazioni,

dei rifiuti, è stato esso stesso fonte d'illegalità. Dallo scorso 30 aprile sono iniziate le iscrizioni al sistema per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno più di 10 dipendenti. Anche sulla base delle informazioni acquisite durante questi primi due mesi di periodo preparatorio, le chiedo quali sono le linee programmatiche del Ministero per correggere le insufficienze e le incombenze del vecchio sistema, soprattutto in considerazione del fatto che la proroga ha avuto proprio lo scopo della revisione del SISTRI. Occorre infatti aggiornare il *software*, introdurre le semplificazioni già segnalate dalle associazioni di categoria, apportare le modifiche sulla base della verifica di funzionamento. Le chiedo inoltre nello specifico se non ritenga pertanto opportuno limitare il sistema ai soli produttori di rifiuti speciali pericolosi, rendere semplice l'utilizzo del SISTRI attraverso regole minime e facili da applicare, esonerare dall'iscrizione le piccole imprese già in sofferenza per la pesante crisi economica e già costrette a subire un forte aumento della pressione fiscale con IMU e TARES. Chiedo infine se sono stati rimborsati i contributi versati negli scorsi anni dai soggetti obbligati, visto che il sistema non è mai partito definitivamente, ovvero se si intendono rimborsare, anche in considerazione della sensibilità dimostrata dal precedente ministro Clini nel sospendere il pagamento di quest'anno. [DE

la ricerca ambientale (ISPRA) nel corso del 2011 che ha evidenziato un grave stato di contaminazione delle acque superficiali di falda nel comprensorio di Malagrotta, dove vi è la discarica più grande d'Italia. Nello studio suddetto si è accertata la presenza di metalli pesanti, di arsenico, di cloro benzene, in concentrazioni notevolmente superiori ai limiti ammessi. Le chiedo quindi, in relazione alla procedura in corso per il reperimento di un nuovo sito per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, se non sia opportuno escludere in via preliminare il comprensorio di Malagrotta Valle Galeria, già così pesantemente pesantemente colpito dai fenomeni di inquinamento derivanti - come lei saprà - non solo dalla discarica, ma anche dell'impianto di raffinazione di idrocarburi. E quindi se non ritenga necessario ed urgente

*(GAL)*. Signora Presidente, signor Ministro, sappiamo che rispetto al 2010 i rifiuti sono diminuiti oggi del 7,7 per cento, scendendo al di sotto di 30 milioni di tonnellate. Qualcuno afferma che la produzione dei rifiuti è scesa a causa della crisi, asserendo che la diminuzione dei consumi ha prodotto, di fatto, anche la diminuzione dei rifiuti. Noi non riteniamo che sia questa che sia questa la motivazione e pensiamo, invece, che siano state le buone pratiche della raccolta porta a porta, della tariffa puntuale e di tutte le altre iniziative che hanno responsabilizzato il cittadino a determinare una riduzione dei rifiuti. Infatti, mediamente, la raccolta differenziata si attesta in Italia

In Calabria e in Sicilia troviamo una situazione a macchia di leopardo, con *performance* disastrose di alcuni territori, cui fanno in contraltare situazioni decisamente eccellenti. Dico questo anche con cognizione di causa, per essere stato fino a pochi mesi fa sindaco di Grammichele, un Comune che ha creduto nella raccolta porta a porta. E crediamo che si può e si deve tendere alla progressiva riduzione dei rifiuti, con risvolti positivi in termini di tutela ambientale e - perché no - di sviluppo, vedi anche le nuove tecnologie. Ecco perché quando parliamo di sostenibilità ambientale non possiamo non sposare la strategia dei rifiuti zero. Siamo a conoscenza di un'ampia attività proveniente da un comitato promotore nazionale per la proposizione di un disegno di legge d'iniziativa popolare perché l'Italia diventi un Paese a rifiuti zero. Si chiede al Ministro se non ritenga di dover istituire un tavolo di confronto

Signora Presidente, signor Ministro, approfitto per sottoporle un problema specifico, ma che coinvolge alcune iniziative imprenditoriali nella mia Provincia. Mi riferisco alle aziende che producono pannolini compostabili, capaci di disgregarsi in meno di 90 giorni, e che lamentano l'impossibilità di commercializzare questo prodotto nonostante la stipula di contratti di vendita con alcuni asili nido non solo della mia Provincia. Questi ecopannolini hanno ottenuto la certificazione di compostabilità, ma il Codice europeo dei rifiuti (CER) a cui fa riferimento il Testo unico in materia ambientale n. 152 del 2006 che regola lo smaltimento dei rifiuti, non contempla ancora la classificazione di tale prodotto per un corretto smaltimento e trattamento. Si chiede se il Ministro in indirizzo, nelle more dell'attribuzione del codice CER egli ecopannolini per un corretto smaltimento e trattamento, non ritenga urgente estendere in maniera provvisoria il codice dell'organico anche al pannolino biodegradabile, onde evitare così il fallimento delle aziende produttrici - alcune purtroppo sono già fallite e, di conseguenza, di scoraggiare probabilmente in maniera irreversibile le iniziative che puntano sull'innovazione del prodotto. È vero che, almeno nella mia Provincia, è stata avviata la sperimentazione in tal senso, ma è chiaro che questa richiede tempi lunghi che potrebbero essere, purtroppo, fatali.

anche in questo caso rispondo, abbastanza schematicamente, provando ad

Gli obiettivi sono naturalmente quelli contenuti nella normativa europea, che dobbiamo recepire anche con l'approvazione della prossima legge comunitaria e trasfondere - e rispondo al senatore Marinello - all'interno del codice ambientale, passaggio

che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana, oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti». La stessa direttiva pone la prevenzione all'apice della gerarchia dei rifiuti, da applicarsi quale ordine di priorità nella normativa della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Non credo che questo possa essere oggetto di discussione. Questa è un'indicazione

centrale non è questo. Il piano sarà presentato in stesura definitiva entro il mese di dicembre.

di legge rifiuti zero. Abbiamo predisposto una consultazione anche con le associazioni imprenditoriali,

infatti, al quale oggi siamo richiamati è la chiusura del ciclo. Anche da questo punto di vista non ho alcuna obiezione a modificare e anticipare gli obiettivi contenuti all'interno della linea di evoluzione che ho descritto. Il problema è riuscire a farlo; il problema è sostenere che oggi, a fronte del superamento di una previsione di un impianto di termodistruzione, c'è un salto di qualità e di quantità nella raccolta differenziata. Questo è ciò che noi dobbiamo provare a fare e questa è l'azione che sto provando a realizzare anche con le Regioni sottoposte a particolari situazioni di crisi e di difficoltà, a partire dalla Campania.

provare a dare delle risposte anche sul fronte dell'impiantistica finalizzata alla prosecuzione del ciclo dopo la raccolta. In molte realtà italiane il problema è che non si realizzano non

anzi, è proposto come alternativa alla realizzazione dei termovalorizzatori. Allora, a mio avviso, come ho detto in più occasioni, proprio chi ritiene che i termovalorizzatori siano una tecnologia superata dovrebbe

dovrebbe essere pacifico che il salto di qualità è possibile e che tutte le autorità competenti possono agire in tale direzione. Sul tema relativo ho disposto che si rinnovi il commissariamento, con alcune specifiche indicazioni: escludere l'utilizzo della Valle Galeria per l'individuazione di un nuovo sito, realizzare un sito alternativo individuando la sede entro il 31 luglio.

Per quanto riguarda il tema SISTRI, vorrei semplicemente ricordare che si tratta di una vicenda incominciata nel 2006

pattuiti, «le riserve sulla non convenienza economica della fornitura, per quanto possano esserci, non saranno mai idonee a inficiare la validità del contratto stipulato, non ricorrendo gli estremi dell'errore essenziale riconoscibile *ex* articoli 1429 e 1431 del codice civile». Perché cito questo elemento? Perché ritengo che sia evidente che l'impalcatura del sistema necessiti di una semplificazione e che, forse, se ci si mettesse oggi a congegnarla, la si ipotizzerebbe del tutto diversa da quella che è stata realizzata. Il punto fondamentale è che noi abbiamo un vincolo di carattere contrattuale,

e facendo in modo che un'eventuale inefficienza del sistema sia causa di una possibile risoluzione del contratto. Voglio dirlo con molta chiarezza: dobbiamo dobbiamo mettere in conto o comunque prevenire il rischio che il sistema non funzioni, ma non possiamo in alcun modo pensare che si superi il principio della tracciabilità dei rifiuti, soprattutto di quelli pericolosi. Quindi, nel momento in cui dovessimo trovarci di fronte al fatto che il sistema non funziona o funziona soltanto parzialmente, dovremmo avere già ipotizzato delle alternative possibili per evitare di rimanere scoperti rispetto alla questione della tracciabilità. Contemporaneamente, dobbiamo produrre una profonda opera di semplificazione delle procedure e anche, naturalmente, di riduzione della platea. Questo è il lavoro che ho iniziato a fare, anche con la costituzione di un tavolo con tutte le associazioni imprenditoriali dato una prima risultanza, ora si tratta di capire in che modo tale risultanza può essere tradotta dal punto di vista normativo e, contemporaneamente, questo è l'altro aspetto,

quello relativo all'adozione del piano nazionale di prevenzione e riduzione dei rifiuti che dovrebbe essere pronto entro la fine dell'anno, quindi tra alcuni mesi, e apprezzo anche il profilo di concretezza che ha voluto dare alle sue affermazioni, andando oltre quello che è stato fino ad oggi troppo spesso un atteggiamento di proclamazione di intendimenti e di scarsa o nessuna concretezza.

Poi, ci dice (è vero come ho detto prima io): se tu non riesci a recuperare la materia, bruciala. Però gli esempi virtuosi italiani, che arrivano al 94 per cento di recupero di materia, ci dimostrano che quel 6 per cento non si brucia, quindi l'incenerimento non

prepariamoci, perché il suo malfunzionamento è già stato dimostrato. Ritengo infatti che tale sistema necessiti di una revisione, a partire da un monitoraggio che permetterà di valutare l'effettiva operatività e applicabilità delle dinamiche attualmente previste, che consentono di contrastare infiltrazioni e illeciti in un ambito già molto contaminato, ma allo stesso tempo evitare che il sistema si trasformi nell'ennesimo labirinto di burocrazia in grado solo di ostacolare le aziende operanti nel settore. Sulle opacità relative alle dinamiche istitutive resto

Ministro, la Lega Nord non è soddisfatta delle sue risposte. Peraltro su alcune domande non è stata data risposta, ma il tempo è tiranno anche per lei. Sulla questione del SISTRI ci sono delle certezze: per errore delle istituzioni hanno già pagato troppo, e forse per nulla, molte imprese, ed altre pagheranno. Pertanto, signor Ministro, la invitiamo ad affrontare questa tematica con efficienza ed efficacia. [DE

non riutilizzabile è composta da pannolini, cicche di sigarette e poco altro. È un problema tecnologico. La tecnologia ci può venire incontro. Allora, facciamo investimenti sulle nuove tecnologie e non sugli inceneritori.